a questa mattina non è ancora pervenuto al Senato il disegno di legge finanziaria e il testo del decreto varato dal Governo la settimana scorsa. ieri pomeriggio è pervenuta la Nota di aggiornamento al DPEF e la Relazione previsionale e programmatica. Nella Nota di aggiornamento al DPEF il Governo registra un incremento di gettito per il 2007, portando il dato di 703 miliardi di euro, tuttora dato ufficiale del bilancio pubblico per quest'anno, a 722 miliardi con un incremento di 19 miliardi di euro per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Noi discutiamo di un assestamento del bilancio dello Stato che - come ho detto la settimana scorsa

euro. Non si capisce, quindi, perché siamo chiamati a discutere ed approvare un assestamento di bilancio per il 2007 che riporta 7 miliardi in meno di quanto il Governo dichiara nella Nota di aggiornamento del DPEF, a parte le mie valutazioni che anche in quella Nota mancano ancora 7-8 miliardi in più di gettito tendenziale per il 2007. Sta di fatto, signor Presidente, che in questo momento

e il decreto predisposto dal Governo la settimana scorsa e non ancora pervenuto al Senato per altri 7 miliardi,

nella Nota di aggiornamento fa emergere 19 miliardi di gettito in più e nel bilancio di assestamento ne indica solo 12.

ricordando, signor Presidente, che, nella settimana passata, le agenzie e i *media* hanno diffuso una dichiarazione

Presidente, questa dichiarazione ha particolare rilievo non soltanto per l'importanza di chi ha pronunciato questa frase, ma anche per la gravità del suo contenuto, una gravità che Senatore Zanda, devo fare una comunicazione su questo punto.

con grande responsabilità di tutte le forze politiche, sul disegno di legge n. 1677 che inerisce agli stessi argomenti e che era fortemente connesso al decreto-legge. La Camera, naturalmente nella sua sovranità, ha compiuto una scelta diversa e le implicazioni, sia di carattere normativo, sia di carattere contenutistico,

sul disegno di legge. Devo quindi riferire che l'8a Commissione, pur convocata questa mattina, ha svolto la discussione generale, ma non si è trovata nelle condizioni di concludere i propri lavori. Per tale ragione, il provvedimento giunge in Aula senza un mandato al relatore. Concludo ricordando che tutti Capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione, nella discussione generale tenutasi stamattina in 8a Commissione, hanno convenuto sulla necessità e l'urgenza di approvare la conversione del decreto‑legge per le sue implicazioni giuridiche e costituzionali, contenendo il testo anche norme di carattere penale. È con tale motivazione che la Commissione ha sostanzialmente rinviato all'Aula il provvedimento.

che il Senato non avrebbe apportato modificazioni al decreto‑legge e che si sarebbe intervenuti sul disegno di legge. Ora abbiamo sentito la senatrice Donati e il rappresentante del Governo, il ministro Bianchi:

per comprendere fino a che punto si è trattato di un incidente tecnico o politico rispetto al testo discusso e approvato dal Senato. Del resto, signor Presidente, abbiamo un problema: ogni volta il Senato dover approvare a scatola chiusa dei provvedimenti con la promessa che alla Camera non succederà nulla, e poi, inevitabilmente (è successo già altre volte in questa legislatura), la Camera si prende dalle licenze; per carità, si dice che nella sua autonomia fa quello che vuole, è l'autonomia che manca a noi. Poiché il Ministro ha affermato in questa sede che il Governo aveva espresso parere contrario rispetto agli emendamenti, e non ho motivo di dubitare della parola del ministro Bianchi, vorremmo capire quali sono le conseguenze di queste modifiche normative. Infatti, signor Ministro, chi ci dà la garanzia che domani riusciremo a mettere a posto le cose, dal momento che lei considera gravi gli emendamenti che sono stati approvati, al punto che il Governo aveva espresso parere contrario? anche per evitare conseguenze negative sulla qualità della legislazione. Quindi, vorremmo sapere su cosa il Ministro è contrario e perché, in modo da essere certi che potremo intervenire con raziocinio quando si dovrà l'esame del disegno di legge. In particolare, vogliamo sapere se è intenzione del Governo prevedere modifiche al disegno di legge attraverso le quali cancellare le norme approvate.

Signor Presidente, intervengo a sostegno delle richieste del senatore Storace. In occasione del passaggio alla Camera, da parte di alcuni esponenti della maggioranza che l'approvazione dell'emendamento su cui il Governo si era espresso in senso contrario era conseguenza di un errore di voto. Quindi, è anche mio interesse sapere se ci troviamo adesso di fronte ad un testo sbagliato

Con questa intenzione si è entrati in Aula, dove però è avvenuto, come ha ricordato ora il senatore Calderoli, che su un emendamento, proposto peraltro da un rappresentante della maggioranza, si sia dato luogo ad un voto di accettazione contro il parere del Governo.

quanto si riteneva che fosse opportuno lasciare intatto il decreto così com'era stato approvato dal Senato, rinviando la discussione nel merito ad una fase successiva. Nel merito, poi, ovviamente il Governo aveva e ha tuttora delle opinioni in parte favorevoli e in parte contrarie agli emendamenti proposti. Gli emendamenti che alla fine sono stati approvati, e che quindi sono contenuti nel testo attuale del decreto, sono sostanzialmente in linea con quanto è emerso dal confronto sia al Senato sia alla Camera. Ricordo, per esempio, che l'emendamento sul quale si è avuto il voto favorevole contro il parere del Governo

(l'ho chiesto ancora stamattina) che il decreto venga approvato così com'è. Gli emendamenti che sono stati apportati al testo del decreto, insieme agli altri che pure erano stati presentati e poi ritirati alla Camera, unitamente a quelli che il Senato intenderà nuovamente proporre saranno oggetto della nostra discussione sul disegno di legge.

creando una Commissione congiunta del Governo, della Camera e del Senato che lavori su un testo condiviso che possa poi essere portato all'approvazione

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti esprime parere non ostativo

il livello di soddisfazione rispetto a questo *iter*, piuttosto travagliato, per cui qui siamo costretti a fare delle cose, alla Camera fanno quello che vogliono, arriva il Governo che ci dice che dalla prossima volta un pezzetto lui, un pezzetto la Camera, un pezzetto il Senato...

Presidente della Commissione quali sono le conseguenze degli emendamenti approvati, nessuno ce l'ha spiegato e credo sia un diritto del Senato deliberare dopo aver conosciuto quello che è avvenuto alla Camera.

che ci viene dalla Camera e che invito tutti a leggere, perché prevede una sanzione per chi tiene il motore acceso allo scopo di tenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. A parte che mi sembra difficile si possa capire, riscontrare, contestare le ragioni per cui, durante una sosta o una fermata, il conducente tenga il motore acceso,

di ferragosto o del periodo estivo sulle nostre autostrade, che dureranno ore e gli automobilisti vivranno nelle loro automobili una sorta di esperienza da forno crematorio, come si può pensare che il comportamento di chi tiene acceso il motore per avere un po' di refrigerio e magari non finire arrostito sia illecito Mi si dirà che, se c'è la coda in autostrada, per fortuna le pattuglie autostradali non potranno passare per elevare le contravvenzioni,

Presidente, l'emendamento introdotto dalla Camera è francamente incomprensibile e io, nel merito, condivido pienamente le osservazioni svolte dal collega Pastore. Pastore. Trovo francamente inaccettabile il comportamento con cui l'altra Camera ha affrontato questo decreto-legge. Siamo stati prima aspramente criticati da autorevoli esponenti della Camera dei deputati per la lentezza con cui abbiamo esaminato il decreto-legge; addirittura c'è stato qualcuno che ha detto che mentre la gente moriva per le strade il Senato discuteva. Viceversa, noi abbiamo esaminato con grande rapidità il testo del decreto- legge

sta parlando di un settore piuttosto importante. Solamente nel settore dell'intrattenimento operano 13.100 dipendenti,

che non sono i divieti rigidi messi rispetto a certi orari che possono determinare la sicurezza sulle nostre strade, ma un insieme di provvedimenti che coinvolga tutti i soggetti, naturalmente a partire dai titolari dei locali. Voglio poi ricordare che l'Aula del Senato, proprio in occasione della discussione sul disegno di legge, ha trovato una diversa soluzione nell'accogliere un emendamento della senatrice Emprin Gilardini, volto a promuovere la sicurezza sulle strade a partire dalla responsabilità

da questo punto di vista, vorrei motivare un voto negativo per senso di responsabilità, pur riconoscendo che nel merito, in effetti, questa norma richiederebbe di essere corretta. Mi auguro che, all'interno del disegno di legge che modifica il decreto-legge, essa venga approvata con quello spirito di sicurezza condivisa e di responsabilità e non invece attraverso inutili proibizionismi che non servirebbero nemmeno a

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Gruppo Insieme con l'Unione-Verdi-Comunisti Italiani voterà questo decreto. Ho già anticipato che lo facciamo responsabilmente perché il Paese ha bisogno di queste norme e non possiamo permetterci di non convertire il decreto-legge in esame in materia di sicurezza stradale. Voglio però ricordare che alcune modifiche introdotte non vedono d'accordo il mio Gruppo e ne voglio citare qualcuna in particolare: le

il tema della sicurezza stradale deve essere un percorso di accompagnamento alla guida e a comportamenti corretti, al di là dell'auto che si può utilizzare.

della nostra Aula. La riduzione a un solo anno fa però venire meno la necessità di un percorso progressivo di addestramento alla guida e di sicurezza stradale. Se veniva spesso invocato il problema delle famiglie

c'è un indebolimento del quadro sanzionatorio, della parte repressiva, da un lato, mentre vi è un accanimento in alcune fasce orarie, Le norme in materia di sicurezza stradale debbono essere ben comprese dai cittadini per essere rispettate. Un'articolazione molto dettagliata di norme che differenziano tra il giorno e la notte non coglie nel segno di un'esigenza di chiarezza nei confronti dei cittadini e delle cittadine, che sono i soggetti tenuti a rispettarle. Peraltro, credo che sia anche molto discutibile sul piano della sicurezza stradale il fatto che tutto ciò che avviene di notte sia gravato da alcune sanzioni, mentre ciò che accade di giorno

Chi conosce i dati sulla sicurezza stradale sa che l'incidentalità ha purtroppo una sua casistica molto drammatica, ma è anche drammaticamente stabile negli orari e nei giorni, nelle località in alcuni fenomeni che avvengono - lo voglio ricordare di nuovo - per due terzi all'interno dell'ambito urbano, proprio perché lì si verifica una concentrazione enorme di traffico e gli utenti della strada sono molteplici. Pensare di introdurre un fondo per l'incidentalità esclusivamente notturna presso la Presidenza del Consiglio non ci sembra un buon servizio alla causa,

non abbia utilizzato né alcool né droga), proprio per garantire la sicurezza di sé e di tutti gli altri utenti della strada, questo deve avvenire all'interno di una cornice in cui si interviene su tutti i soggetti responsabilmente in un quadro integrato con campagne mirate. Separare invece questo tema dal Ministero dei trasporti, dedicarvi delle risorse specifiche, portarlo presso la Presidenza del Consiglio ci sembra un modo un po' inutile e fuorviante di disgregare e di mal utilizzare delle risorse. Ripeto, sì a campagne mirate e no a un fondo istituito fuori dal Ministero dei trasporti

Presidente, il Senato, con grande senso di responsabilità, aveva approvato contemporaneamente entrambi i provvedimenti - sia il decreto-legge che il disegno di legge -, affinché gli stessi potessero essere esaminati insieme alla Camera, in quanto fortemente collegati. Sappiamo che questo poi non è avvenuto ed oggi ci ritroviamo nuovamente a discutere ed ad approvare, con molta fretta, dati i ristretti tempi di conversione, il solo decreto-legge, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati. È evidente come non sia possibile procedere ad un esame organico della normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale, anche perché il disegno di legge, approvato nelle scorse settimane, ha subito modifiche anche sulle norme che sono poi riprodotte nel decreto-legge, a sua volta modificato dalla Camera. Ciò crea una profonda confusione che mette seriamente a rischio la possibilità di adottare efficaci iniziative per contrastare l'elevato numero di incidenti sulle nostre strade. Entrando nel merito del decreto-legge, esso riproduce in materia di sicurezza stradale gli stessi nodi problematici che sono stati posti all'attenzione dell'Assemblea durante l'esame del disegno di legge. Ciò fa pensare che non esista una reale volontà del Governo di adottare concrete iniziative volte a contrastare il grave fenomeno degli incidenti stradali nel nostro Paese. Infatti, analizzando il testo, si osserva che esso in realtà è fortemente indirizzato all'adozione di diverse misure che hanno, in primo luogo, una natura sanzionatoria, lasciando un ridotto spazio a quelle iniziative di natura preventiva che hanno avuto, invece, ampio riscontro durante l'esame del citato disegno di legge. Il Governo, ad esempio, al fine di contrastare il numero di morti e feriti che ogni anno si registrano sulle nostre strade, non ha ritenuto urgente e necessario attuare un immediato intervento sull'ammodernamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture, sul miglioramento della segnaletica stradale oppure sul potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Sono iniziative, queste, dalle quali non è possibile prescindere ai fini dell'attuazione di una concreta iniziativa in materia di sicurezza stradale. Tuttavia, riteniamo che le problematiche che interessano la sicurezza stradale siano state affrontate nel decreto-legge in maniera soltanto parziale ed è per questo motivo che chiediamo alla maggioranza e al Governo, nell'ambito dei prossimi interventi in materia, di adottare, con maggior coraggio e determinazione, iniziative concrete volte a rendere la circolazione sulle strade più sicura, a tutela della vita dei cittadini.

deputati non ha avuto modo di approvare il disegno di legge, come era in parte previsto dal precedente passaggio in Senato,

Le modifiche non sono tutte convincenti. Ne accennerò essenzialmente due: la prima riguarda la diminuzione da tre ad un anno del periodo in cui il neopatentato non può guidare auto di una certa potenza.

con la conseguenza di escludere le famiglie meno abbienti da questa possibilità, proprio quelle famiglie per cui la patente costituisce

del neopatentato che non sulle possibilità di guidare certe autovetture. Oltretutto, l'aumento del patrimonio circolante di per sé costituisce un

di veicoli circolanti estremamente maggiore di quella che sono in grado di sopportare. Quindi, immettendo ulteriori autovetture nel circuito non facciamo altro che peggiorare il livello di sicurezza stradale, escludendo peraltro proprio

durante una sosta o una fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento: è di per sé un uso sbagliato

era tutto orientato sull'incremento dei controlli, delle pattuglie e così via. Oltretutto, i limiti che oggi si incontrano in ordine all'ampliamento dell'educazione stradale nelle scuole sono più legati alle possibilità di coordinamento e di intervento del Ministero dei trasporti sui programmi scolastici, che non a un *deficit* di risorse in questo ambito. Complessivamente, quindi, il decreto non è mutato nelle sue tratte essenziali dal passaggio alla Camera; pertanto, il nostro Gruppo mantiene la posizione di astensione che lo aveva caratterizzato già nel precedente passaggio Signor Presidente, come era prevedibile (il signor Ministro lo sa perché ne abbiamo parlato questa mattina in Commissione), alla Camera sono stati meno indulgenti e hanno sostanzialmente modificato (è inutile nascondersi dietro ad un dito, perché il testo è stato sostanzialmente modificato) quanto partorito dal Senato, con fatica e con fiducia nei confronti del Governo. Non Non sfugge a nessuno il fatto che il via alle modifiche del testo, così come onestamente il Ministro ha affermato anche durante il dibattito in Commissione, sia stato dato dalla sua stessa maggioranza, per cui, una volta modificato il testo, la Camera ha pensato di migliorarlo sostanzialmente. Ciò significa però che anche sulla questione della sicurezza stradale siamo al cospetto di una maggioranza che manifesta tutte le fratture politiche possibili e immaginabili. Del resto, come le ho detto, signor Ministro, l'imboscata della sua maggioranza, che era un dispettuccio a lei, non personale ma in quanto rappresentante del Governo,

che proprio in Commissione trasporti avevamo inaugurato, consentendole di proporci un nuovo strumento legislativo, quello del cosiddetto decreto a perdere. Non credo che in futuro ci sarà da parte di questa minoranza, quantomeno da parte del di AN, la medesima comprensione nei confronti del Governo. Anche la strada da lei tracciata relativamente alla possibilità, che potrebbe essere anche un esempio di buon senso, di mettere insieme quanto di buono emerge dal confronto tra il Governo, la maggioranza e la minoranza, sia alla Camera che al Senato, costituisce uno strumento nuovo al quale guardiamo con sostanziale diffidenza proprio in virtù di quanto accaduto accaduto in questi giorni. Cosa resta allora sul tavolo politico? Resta l'evidente schizofrenia legislativa di un disegno di legge che si sovrappone ad un decreto e di un decreto che si sovrappone a un disegno di legge; resta il nostro ragionamento, che Alleanza Nazionale ha posto all'attenzione politica sin dall'inizio (cioè, dal nostro punto di vista occorreva dare più spazio alla prevenzione, all'educazione e alla formazione, piuttosto che alla repressione fine a se stessa e alle sanzioni per far cassa); resta anche il fatto che molte delle proposte avanzate da Alleanza Nazionale e bocciate in Senato disegno di legge alla Camera, migliorando sostanzialmente il testo, che comunque dal nostro punto di vista resta carente. Avevamo parlato del fondo sull'incidentalità notturna, che è stato poi puntualmente inserito nel testo alla Camera grazie ad un emendamento di Alleanza Nazionale, che di fatto dota il Governo delle risorse necessarie per intervenire affrontando dignitosamente questo fenomeno. Avevamo parlato del divieto di somministrare le bevande alcoliche dopo le due di notte, uno squarcio nell'ipocrisia della tabellina sui rischi derivanti dall'assunzione di alcol prima di mettersi alla guida, che avrebbero dovuto affiggere i gestori e i proprietari di locali notturni,

dal ragionamento proposto da qualche collega che mi ha preceduto perché crediamo che dalle due in poi nei locali notturni si possa comunque bere, si possano comunque somministrare

alla velocità - come dicevamo poco fa - il provvedimento è stato modificato. Certo poi ci sono anche delle sciocchezze, come quella che ha rilevato il senatore Pastore all'articolo 3-*bis* in materia di accensione del motore durante la sosta del veicolo. Quella è veramente una sciocchezza. allora il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà? Si asterrà dalla votazione perché, come abbiamo detto anche in Commissione, siamo consapevoli di non poter beneficiare di altri 8‑10 passaggi parlamentari per migliorare ulteriormente questo provvedimento; si asterrà perché questo Governo non ha una politica né sulla sicurezza della strada, né sui trasporti; si asterrà perché la sicurezza non si introduce e si salvaguarda solo con le sanzioni e con la repressione ma anche con i controlli preventivi, con l'educazione e con la formazione.

FANTOLA *(UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che ci saremmo potuti aspettare di tutto in questa travagliata legislatura ma non l'alt della Camera dei deputati a questo provvedimento sulla sicurezza stradale; un alt imposto dalla Camera, peraltro a poche ore dalla sua scadenza. Nell'altro ramo del Parlamento la maggioranza, come ha riconosciuto ed affermato con sincerità il Ministro in Commissione, si è spaccata; il Governo è stato battuto su un provvedimento sul quale qui in Senato l'opposizione aveva assunto un atteggiamento serio, aperto al dialogo, vorrei dire persino di sostanziale condivisione del provvedimento stesso. Un atteggiamento testimoniato dal lavoro di approfondimento del testo svolto in Commissione e in Aula e dalla condivisione della mia parte politica, ma anche delle altre parti politiche di minoranza, di minoranza, di un percorso di decretazione d'urgenza per far sì che alcune norme entrassero in vigore in un momento critico, prima dell'estate, che alcune norme tese ad elevare il livello di sicurezza stradale

che la dichiarata incapacità e impossibilità della maggioranza di approvare l'intero disegno di legge alla Camera dei deputati e al Senato prima della scadenza dei termini del decreto

Ma è evidente a tutti che la nostra astensione rappresenta un segnale di grande attenzione per il tema, per il provvedimento, per le disposizioni contenute nel provvedimento, per l'*iter* e per il clima con il quale è stato affrontato il tema della sicurezza stradale.

che proprio alla Camera, dove ha una maggioranza se non bulgara sicuramente ampia, non risulta tale al momento del voto. Ma ciò non è così, perché è un problema che interessa tutta l'Aula,

decada al Senato se non è approvato entro oggi, con conseguenze gravi in materia di sicurezza dovute al vuoto normativo che ne deriverebbe. Pensate che verrebbe sostanzialmente sostanzialmente annullata la pena per chi guida senza patente o per chi si rifiuta di sottoporsi alle prove dell'alcolimetro o sull'uso di stupefacenti.

come la maggiore attenzione alla formazione continua nelle scuole, l'istituzione di un fondo di contrasto per l'incidentistica, l'interruzione delle vendite degli alcolici dopo

Di fronte ad un'opinione pubblica che chiede una risposta chiara, netta e forte

collega di Gruppo, ma non arrivo alla stessa conclusione. Questo è un provvedimento che non ritengo assolutamente atto a fornire le risposte che i nostri cittadini si aspettano; anzi, è espressione di una minoranza del Paese che cerca di risolvere alcuni problemi,

il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore del provvedimento di conversione essenzialmente per senso di responsabilità istituzionale. Nella presentazione al disegno di legge sulla sicurezza stradale, approvato da quest'Aula appena due settimane or sono, in qualità di relatore non feci velo di un significativo ruolo esercitato dall'opposizione, che in un dibattito costruttivo, non facile, con la maggioranza e il Governo aveva saputo dare, pur nella differenza di ispirazione culturale, di analisi e di strategia, il suo significativo contributo, in alcuni casi, a mio avviso, anche migliorando il provvedimento finale.

Allo stesso modo sono rimasto e rimango sorpreso dell'esito della discussione alla Camera. Non ritengo sia il caso di alimentare purtroppo non anacronistiche contrapposizioni o diatribe istituzionali, ma è certo che l'esito di quella discussione ha rischiato di creare grave pregiudizio non al Governo (cui va dato atto, in particolare al Ministro, di essersi speso totalmente per l'approvazione di questo provvedimento), ma a quei cittadini che negli ultimi mesi sono incorsi in sanzioni penali e amministrative e soprattutto a quelle attività commerciali che rischiano di essere gravemente danneggiate dal provvedimento in approvazione. Ciò che ne risulta è uno stato di incertezza e di indecisione normativa che genera soltanto ulteriore discredito dell'opinione pubblica nei confronti di chi è chiamato a rappresentarla nelle massime istituzioni dello Stato. Non voglia questa mia riflessione sembrare una censura alle prerogative dell'altra Camera, ma certo è che altro poteva essere il comportamento di assoluto buon senso, vale a dire, in pratica, la ratifica della legge di conversione del decreto‑legge così come licenziata dal Governo, come del resto, non senza qualche sofferenza e disappunto, ha fatto quest'Aula per concentrarsi doverosamente sul disegno di legge, anche in vista (poteva essere naturale prevederlo) di eventuali modifiche in terza lettura. Centrale per noi rimane l'approvazione del disegno di legge. Si rende pertanto indispensabile una qualche forma di coordinamento maggiore tra le due Camere e in modo particolare tra le due Commissioni, onde evitare il pendolo della navetta. Nel merito del provvedimento, è doveroso - assolutamente doveroso - rilevare come le modifiche apportate dal centro‑destra alla Camera non siano marginali. Esse in un certo stravolgono le disposizioni di legge e probabilmente in certi casi vanno ben oltre il limite e il merito della materia della sicurezza stradale. Mi riferisco segnatamente alla modifica all'articolo 6

aggiungere che l'articolo 6-*ter*, in maniera assolutamente demagogica, destina e vincola le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative, come veniva ricordato anche nell'intervento della senatrice Donati, a corsi di educazione stradale. Probabilmente, conformemente a come questa

senatore Pecoraro Scanio. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, è necessario, in premessa, sottolineare come il provvedimento che oggi discutiamo, nella sua formulazione trasmessa dalla Camera a questo ramo del Parlamento, fosse un testo estremamente problematico. Problematico sotto diversi profili: nei princìpi che lo ispiravano, in materia di competenze dei diversi organi costituzionali, nella scarsa ambizione in esso contenuto. Si trattava di un testo fortemente ideologico che avrebbe messo in discussione la capacità di programmazione del territorio da parte degli enti locali. Questa è la prima riserva che abbiamo posto a quel testo pervenuto alla discussione della Commissione: ritenere che la programmazione del territorio da parte degli enti locali sia solo un impiccio di fronte alle aspettative dell'impresa è sbagliato, profondamente sbagliato. L'equilibrio tra l'interesse pubblico e le convenienze del singolo non deve essere compromesso e la prevalenza degli interessi di tutti deve sempre avere un valore superiore. Troppo spesso assistiamo a sindaci che, in nome dello sviluppo, accettano di mettere in discussione questo principio. Se negli anni Ottanta il debito era la leva per garantire sviluppo e coesione sociale, oggi in tante città il consumo del territorio ha sostituito il debito: costruzioni abusive tollerate, piani regolatori e varianti dal mattone facile, scempi addirittura nelle aree protette. Queste situazioni sono sotto gli occhi di tutti e soggiogare la volontà di una assemblea democraticamente eletta

all'impresa che certifica, si è rischiato di aprire un fronte di contenzioso perenne tra pubblico e privato: si prevedeva che l'amministrazione nel solo atto di ricevere la domanda acconsentisse all'avvio dei lavori e delle attività, senza neppure verificare cosa contenesse quella domanda, se le prescritte certificazioni o una risma di fogli bianchi. Non si tratta di stereotipato antisviluppismo, ma di mettere in discussione la qualità dello sviluppo stesso. Dal punto di vista costituzionale, dimenticare l'articolo 117 e avocare allo Stato centrale tante e tali competenze avrebbe messo in discussione l'equilibrio tra Regioni e Stato centrale stesso. Non basta scrivere al primo comma del primo articolo di una legge che essa riguarda i livelli essenziali di prestazione perché venga meno il conflitto tra i livelli sussidiari e una norma di questo tipo, senza neppure un riferimento all'ordinamento regionale, sarebbe stata palesemente incostituzionale. Infine, e questa purtroppo è stata una riflessione che non è riuscita ancora a permeare neppure i lavori del Senato, non possiamo tacere la scarsa ambizione di questo provvedimento. La nostra economia sta sempre più diventando immateriale e cognitiva: non si producono più merci, ma idee. È un cammino ancora lungo, ma che è iniziato e che deve essere accompagnato: prevedere una uguale normativa per l'industria pesante e che consuma territorio e per le imprese cognitive e dei servizi è un'occasione perduta, che non solo immobilizza una realtà in mutamento, ma rafforza i cambiamenti climatici in corso, che tutta quest'Aula pochi mesi fa ha ritenuto essere uno degli elementi di maggiore allarme che ci si para davanti. Questo era il contesto che la Commissione si è trovata davanti e devo dare atto della sensibilità dei colleghi e del Governo nel recepire alcune di queste istanze e nel modificare radicalmente l'impostazione originaria del provvedimento: sono stati infatti introdotti alcuni correttivi sostanziali. Permane la precedente normativa nel caso che una domanda sia in contrasto con il piano regolatore, e quindi la domanda viene rigettata, a meno di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Se l'impresa ottiene il cambio di destinazione dell'area, deve operare per almeno cinque anni, mettendo così un freno alla speculazione edilizia. La consegna della domanda allo sportello unico non dà più diritto all'avvio delle attività, ma consente all'Amministrazione almeno venti giorni di tempo per verificare la documentazione. Sono esclusi da questa normativa i servizi di telecomunicazione e i centri commerciali. Sono, questi, elementi qualificanti del testo alla discussione dell'Assemblea che vanno sottolineati con forza, pur rimanendo alcuni elementi negativi, come il termine perentorio perché il Consiglio comunale valuti le varianti, o la reintroduzione dì previgenti norme relative alla Conferenza dei servizi in un quadro costituzionale ormai mutato. La direzione intrapresa dalla Commissione rimette comunque in equilibrio l'interesse pubblico e l'interesse privato: ci auguriamo che questa direzione sia confermata dall'Aula; ovviamente, sullo stesso indirizzo, si può ancora migliorare. In questo senso poniamo all'attenzione dell'Assemblea alcuni punti che riteniamo qualificanti. Il più rilevante è che, nel caso sia previsto il permesso di costruire, sia prevista ancora la Conferenza dei servizi. Come è noto, la potestà regionale è titolata a decidere in quali situazioni sia necessaria la DIA e in quali sia utile una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, con il rilascio del permesso di costruire, tranne alcuni casi minimi, come la costruzione di nuovi edifici. Noi rischiamo di annullare questa potestà e addirittura di ritrovarci con nuovi fabbricati commerciali o industriali, come alberghi e capannoni, senza che il Comune e la Regione possano svolgere la propria funzione di programmazione, e questo nonostante i venti giorni introdotti al comma 15. E' un punto rilevante per il quale proponiamo con gli emendamenti una soluzione ragionevole. L'altra incognita riguarda la nuova conferenza dei servizi telematica, sulla quale concordiamo che debba essere fatto un investimento, ma d'altro canto è necessaria la giusta gradualità. Limitare le modalità di tale procedura, senza prevedere l'uso, per esempio, della posta elettronica certificata, rischia di svuotare questo importante processo di informatizzazione. Queste sono alcune delle proposte di merito che avanziamo per concludere il cammino iniziato in Commissione. Siamo convinti che in questa occasione il bicameralismo abbia dato buona prova, evitando, se il provvedimento non verrà stravolto dall'Assemblea, che una cattiva legge entrasse nell'ordinamento, ma non possiamo non sottolineare come a tutt'oggi, di fronte ai tanti provvedimenti in questo momento all'attenzione dell'Aula, questo non fosse sicuramente il più urgente.

direttamente a lei, ma all'ufficio in assoluto - cercherà di trovare una giustificazione ad un fatto che, a mio avviso, resta assolutamente ingiustificabile e inqualificabile. Stiamo svendendo la credibilità

interessato e preoccupato, come credo la maggioranza dei senatori e delle senatrici. Quindi, se vogliamo suddividere il suo ragionamento in due aspetti, c'è n'è uno, più generale, che riguarda

coloro che sostengono la semplificazione delle pratiche di avvio e di gestione delle imprese e chi crede ancora nella sburocratizzazione, nonostante le fossilizzate strutture della pubblica amministrazione. Si tratta di un'iniziativa parlamentare e, quindi, non si può non esprimere rammarico per l'occasione mancata ancora una volta da parte del Governo, che, come sembra preferisca fare, ama rincorrere le riforme anziché anticiparle e prevenirle con delle proposte risolutive. Uno dei problemi più fastidiosi per chi intende aprire un'impresa oggi in Italia è rappresentato dalla lungaggine delle procedure e dalla complessità della documentazione da presentare. Molti, infatti, cominciano il percorso, poi si scoraggiano e lo lasciano a metà. Questo vale soprattutto per le imprese familiari e per le piccole e medie imprese, per le quali la burocrazia costituisce un costo suppletivo, spesso insostenibile. Ben venga, quindi, questa legge che in venti giorni, almeno sulla carta, potrebbe consentire di partire con un'attività imprenditoriale.

qualche strumento in più a chi intende accettare la sfida o almeno provarci. Penso soprattutto ai giovani, i quali, solitamente con pochi mezzi a disposizione, sono i primi ad abbandonare, scoraggiati, di fronte agli ostacoli procedurali,

di questa norma, che va concordata e presentata anche a coloro che vivono dall'altra parte dello sportello, c'è forse la difficoltà nel farla passare in tempi rapidi su tutto il territorio nazionale. Questo provvedimento va nella giusta direzione, perché responsabilizza nella stessa misura sia il privato, che lancia la sua sfida, sia la pubblica amministrazione, che la deve accettare sulla base delle nuove regole.

L'autocertifìcazione e l'autodenuncia di inizio attività dovranno diventare prassi consolidata e normale nel rapporto pubblico-privato, con un accentuato livello di responsabilizzazione soggettiva. Tale nuovo rapporto intende favorire la trasparenza e la sicurezza, garantite da un sistema di controlli sia preventivi che successivi da parte della pubblica amministrazione in un confronto diretto con l'interessato. Verrà ridotto anche quel tasso di conflittualità permanente che ha caratterizzato, finora, il rapporto tra l'imprenditore e la pubblica amministrazione, quella diffidenza che spesso ha reso pessimi servizi anche all'efficienza.

pubblica, questa legge sembra avere trovato l'equilibrio per tutelare la presenza dell'iniziativa privata senza dispersione di risorse e con pregevole concretezza. Ora bisogna verificare se alla teoria corrisponderà davvero la pratica, cioè se la legge sarà applicata nel rispetto dello spirito con cui è stata portata fino alla sua approvazione. sua approvazione. Occorre attivare soprattutto gli addetti ai lavori, quelli che stanno dall'altra parte dello sportello, rispetto al fruitore, al cittadino. Il nostro Gruppo ha avanzato alcune proposte emendative che hanno lo scopo di accorciare i tempi dell'attesa di taluni passaggi e di rendere più certi i termini di altri, senza che siano affidati a fumose e prudenziali formule attendistiche indefinite. Resta da verificare se il provvedimento accontenti tutti, e comunque se le esigenze collegate alle diverse zone produttive del Paese trovino pratiche possibilità di adattare il provvedimento stesso alle proprie particolarità. Penso soprattutto alle zone sensibili e, ancora una volta, mi vengono in mente le zone di montagna. In questo caso va detto che proprio nelle zone di montagna vi è stata recentemente una sperimentazione, che potrebbe tornare utile al Governo, di sportello unico. Vorrei ricordare che quando, in ogni circostanza possibile, si parla di montagna e della sua specificità, non si fa un esercizio di presunzione o di pretesa di avere privilegi o trattamenti particolari; ma la montagna non è riconducibile ad un settore generalizzato o tanto meno ad una materia generica. La montagna è un sistema a sé stante; lo dice l'articolo 44 della Costituzione: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Quindi, anche in questo caso, con un provvedimento che può avere, se realizzato nel suo spirito, una presa popolare molto forte, occorre che esso vada garantito a tutti, anche a coloro che abitano in zone problematiche come la montagna. Dicevo che vi è stato un esperimento, proposto dall'UNCEM (l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), di uno sportello integrato; un esperimento effettuato nella zona del Cadore con buoni risultati di operatività concreta sul territorio, tant'è che subito dopo, nel biennio 2002-2003, l'UNCEM ha portato avanti ancora una volta il processo con "*e-Mountain*", un modello tecnologico per lo sportello unico, su addirittura cantieri sperimentali sul territorio nazionale. Questo per arrivare alla definizione di un modello organizzativo, operativo e innovativo trasferibile a tutti i territori montani. Vi sono tratti comuni di questi cantieri, quali il coinvolgimento dei Comuni e di tutti gli altri attori territoriali, la gestione in forma associata dei servizi e l'utilizzo di Internet per mantenere e facilitare la comunicazione. Proprio sull'utilizzo di Internet e sugli aspetti tecnologici questo modello ha incontrato alcune difficoltà. Insomma, anche in questo caso, signor Sottosegretario, prima di costruire le famose cattedrali nel deserto, prevedere qualche misura particolare non sarebbe male: le famose misure compensative dei prevedibili, maggiori costi per determinate località. di montagna perché questa è l'espressione dalla quale pervengo, ma penso con altrettanta preoccupazione alle zone costiere e alle zone meno favorite in genere. Ecco che allora, facendo tesoro di queste sperimentazioni, in qualche caso si deve prendere atto della non giustificabilità di certi costi di attivazione di fronte ad un numero di pratiche che rimane fatalmente basso rispetto a quanto può accadere nelle grandi città. Questo volume di pratiche rende anche economicamente poco sostenibile e organizzativamente complessa l'apertura di uno sportello *ad hoc*; quindi, anche in questo disegno di legge occorre prevedere che che requisiti fondamentali non debbano essere la economicità e la remuneratività dello sportello, ma privilegiare l'aspetto di servizio, il significato di servizio comune e sociale che esso deve avere. C'è poi un tema importante: la difficoltà nel coinvolgere molte amministrazioni extracomunali accanto a quelle comunali. Ecco allora che c'è una proposta concreta che emerge dall'esperienza fatta da UNCEM, quella di ufficializzare e di rendere legale il meccanismo di in modo che quando manchino delle amministrazioni rilevanti si abbia comunque la possibilità di procedere con delle decisioni. Altro meccanismo importante che ho citato prima è quello della autocertificazione,

Anche l'obbligo, da parte di chi fornisce un servizio, di rendere visibile lo stato di avanzamento e gli esiti dei procedimenti via *web* è risultato un appesantimento economico ed operativo inutile e ingiustificato, soprattutto in aree dove non esiste una copertura della banda larga, pertanto prive sia di una domanda di servizi *on line*, sia della fattiva possibilità, da parte di chi deve dare risposte, di fornirle, perché non c'è il collegamento. Si è quindi comprata la frusta prima del cavallo, come si usa dire, almeno in determinate circostanze. Una delle condizioni per cui la trasmissione di un documento elettronico, quindi l'avvio di un reale rapporto *web*, attraverso i miracoli che l'informatica ci fornisce, è di garantire a tutti la possibilità di accesso ai collegamenti, soprattutto per quelle pratiche che hanno un valore legale. Ciò può avvenire anche attraverso un sistema pubblico di connettività. Questa rete però non sarà disponibile - lo sappiamo - in larga parte del Paese ancora per un bel po' di tempo. A questo punto il Governo deve porsi il quesito di come procedere per non creare, all'interno di un medesimo Stato, cittadini di serie A, forniti di banda larga e di tutte le possibilità di collegamento *on line,* e cittadini di serie B, ossia coloro che, in virtù di difficoltà ambientali e di collegamento, non avranno queste *chance*. Il primo provvedimento che emerge da questa esperienza realizzata in montagna, utile anche nelle altre località, è di preparare professionalmente il personale per questo nuovo sistema di contatto con il privato. Il secondo provvedimento, di carattere tecnologico, è di procedere al cablaggio informatico, globale, su tutto il Paese e quindi anche per le zone di montagna e per le zone che hanno altri motivi di svantaggio. Tutto questo, signor Presidente, Sottosegretario, potrà consentirci di guardare con effettivo ottimismo e con accenti positivi, come quelli con cui ho aperto il mio intervento, anche all'apertura di questo sportello unico. Non deludiamo i cittadini dopo questo segnale positivo e dopo questa riforma molto attesa di sburocratizzazione, di semplificazione, di apertura verso l'efficienza e la trasparenza. Sarebbe davvero un guaio a questo punto compiere anche un piccolo costituirebbe un atto di sfiducia non solo verso il Governo, ma verso tutti noi. Come può notare, Sottosegretario, anche dai banchi dell'opposizione siamo pronti a dare il nostro sostegno perché questa legge venga

Signor Presidente, colleghi senatori, la legge posta oggi in discussione prevede lo snellimento delle procedure attinenti lo sportello unico per le attività produttive. Anche questo provvedimento quindi, pur non rientrando tra quella tipologia di norme che abbatte steccati al libero esercizio delle professioni, si inserisce, per le finalità che persegue, nella tipologia di quei provvedimenti legislativi che consentono lo sviluppo e facilitano lo sviluppo imprenditoriale attraverso lo snellimento delle procedure. È fuori dubbio che un provvedimento con questi scopi va ad impattare con una serie di questioni di diritto e di tutela del territorio che devono essere salvaguardate, perché poste a garanzia della comunità, compresa quella imprenditoriale. Ci si è quindi trovati di fronte alla necessità di non limitare le autonomie degli enti locali, che sono garantite dalla Costituzione, e alla necessità di non stravolgere la legge n. 241 del 1990 sulla semplificazione amministrativa (legge non sovraordinata alla presente legge, ma legge di princìpi) e infine dalla necessità di accorciare troppo i tempi della procedura, la cui eccessiva brevità potrebbe impedire una ponderata valutazione delle condizioni sia da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, sia alle imprese richiedenti, che potrebbero esporre i propri investimenti in attività non autorizzabili. Tutte queste osservazioni sul testo licenziato dalla Camera sono state puntualmente evidenziate dalla 1a Commissione permanente e dalla Commissione ambiente e territorio e la 10a Commissione ha fatto in modo di recepirle. Ciò ha portato ad una profonda modifica del testo licenziato dalla Camera, senza peraltro stravolgere lo scopo di semplificare le procedure che l'articolato si poneva. Le novità più consistenti sono state introdotte nei commi 9, 13, 14 e 15 dell'articolo 1, i quali consentono, a chi voglia realizzare o modificare un impianto produttivo, l'avvio dei lavori solo dopo 20 giorni dalla presentazione allo sportello unico di una dichiarazione attestante la sussistenza degli specifici requisiti previsti dalla legge per la realizzazione di quell'opera, corredata dal progetto e da una dichiarazione di conformità alla normativa applicabile, in particolare sugli aspetti edilizi, urbanistici, alle norme igenico-sanitarie e in materia di sicurezza, rilasciata dal progettista sotto la propria responsabilità. La Commissione, in particolare, per arrivare al testo presentato, ha cercato di tutelare maggiormente le parti interessate, modificando in due punti il testo licenziato dalla Camera: al comma 13 è stato introdotto l'obbligo per il progettista di munirsi, oltre che dell'idonea assicurazione per la responsabilità professionale, anche di quella per l'ammontare del valore dell'opera e, al comma 15, il termine dei 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione e la contestuale ricevuta, quale titolo autorizzatorio, da parte dello sportello unico, prima dell'avvio dei lavori, al fine di consentire le verifiche necessarie da parte dell'ente locale. Per chi conosce i tempi di risposta della pubblica amministrazione, specie di quegli enti locali che hanno maggiori dimensioni, sa perfettamente che 20 giorni sono un'inezia per attivare una procedura di verifica e, probabilmente, il rispetto di questi tempi li metterà a dura prova nella loro organizzazione, se si tiene conto che molti Comuni sono sotto organico. Tuttavia, si è voluto dare un segnale chiaro: chiedere alla pubblica amministrazione di organizzare meglio le proprie risorse e rispondere in tempi certi e ragionevoli alle istanze dei cittadini. Il tempo d'attesa prima dell'inizio lavori permette un controllo ancora in fase di dichiarazione, non previsto dal testo licenziato dalla Camera, perché si sa che la messa in pristino (pur essendo prevista dalla presente legge negli articoli successivi), richiede una procedura molto complicata e, soprattutto, risulta onerosa per gli imprenditori, sia perché è a loro carico, sia perché comporta spreco di tempo per investimenti non fattibili. L'abbreviazione dei tempi per le singole procedure previste è una costante di questa legge. Così, se presentata la dichiarazione occorrono chiarimenti sulle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, chiunque sia interessato (lo sportello unico d'ufficio, il richiedente, le associazioni o i comitati) convoca una riunione entro tre giorni, anche nel caso in cui non sia possibile, per la tipologia dell'intervento rientrante, di cui viene redatto verbale che vincola le parti, senza che ciò interrompa le attività già avviate. Inoltre, qualora la tipologia d'intervento non consenta la sua attivazione immediata, perché rientra nella casistica individuata all'articolo 2, ricevuta la domanda di autorizzazione, lo sportello unico deve convocare la prima riunione della conferenza di servizio entro sette giorni dalla presentazione della domanda e il verbale conclusivo della conferenza deve essere perfezionato perfezionato e comunicato entro i successivi 30 giorni. Anche in questo caso, se non vi sono motivi di dissenso espressi nel verbale, le opere possono iniziare immediatamente. Anche questa è una modifica della procedura indicata dalla legge n. 241 del 1990, atta a favorire l'impresa sia per la rapidità dei tempi che per lo snellimento dell'*iter*. spirito si ritrova anche nel mettere a norma la procedura in caso di dissenso da parte degli amministratori coinvolti nel procedimento, perché la legge ora in esame pone vincoli temporali al Consiglio dei ministri, qualora l'amministrazione procedente o dissenziente sia statale, ovvero agli organi esecutivi di Regione, Provincia e Comune negli altri casi, i quali devono assumere una decisione al massimo entro 75 giorni. Tempi certi, il cui mancato rispetto può essere passibile di ricorso da parte dell'imprenditore. Ovviamente, ritenendo giusto seguire i suggerimenti della 1a Commissione di salvaguardare le esperienze già maturate dagli sportelli unici di molti Comuni, qualora il progetto di impianto produttivo non risulti conforme agli strumenti urbanistici, viene rigettato dal responsabile dello sportello unico. Credo che questo punto costituisca un nodo importante,

Con questa legge viene dato spazio e responsabilità ai tecnici professionisti: oltre alla dichiarazione iniziale anche il collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. I controlli sono sempre attivabili, così come l'adozione delle misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che devono essere comunicate allo sportello unico e all'interessato, che può chiedere attivazione alla conferenza dei servizi. Se si accerta che sono state rese dichiarazioni o autocertificazioni false, queste sono trasmesse alla competente procura della Repubblica. Sui controlli merita spendere ancora qualche parola perché vengono sollecitate azioni sinergiche attraverso stipulazioni di intese tra prefetture, uffici finanziari competenti per territorio e tutte le amministrazioni competenti per definire modalità e criteri per l'esecuzione dei controlli

le riunioni di chiarimento e soprattutto su cui è possibile conoscere ad ogni momento le informazioni sulle dichiarazioni, sulle domande presentate, sul loro *iter* procedurale e sugli atti adottati anche in sede di controllo successivo. Questo sarà possibile perché lo sportello unico è obbligato a mettere in rete, senza ledere il diritto alla riservatezza, come esplicitato al comma 6 dell'articolo 1, senza indugio e gratuitamente tutte le informazioni che prima citavo. Quindi, l'imprenditore, ma anche tutti gli altri soggetti interessati, beneficiano di informazione e trasparenza da parte della pubblica amministrazione. Per questa ragione la conferenza di servizio è pubblica e vi possono partecipare senza diritto di voto i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, che però possono proporre osservazioni. È quindi questa una una legge atta a portare fiducia agli imprenditori per incrementare le loro attività produttive, facilitando le procedure per dare avvio ai lavori, assegnando a ciascun attore del procedimento la responsabilità che gli compete, garantendo così i molteplici interessi presenti sul territorio. Auspico infine che nel corso della discussione si possa ulteriormente migliorare l'impianto della legge, accogliendo alcuni emendamenti che meglio puntualizzano e garantiscono un *iter* e una gestione corretta, garantendo diritto e certezza dei tempi, ma anche tutela dell'ambiente e del territorio.

transitare un disegno di legge, già approvato dalla Camera, che interviene in maniera anche significativa sul rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, tra pubblica amministrazione ed in particolare le imprese, rappresenta una novità nel panorama di questa legislatura che, al di là di qualche affermazione di principio, non ha mai visto in maniera seria discutere e deliberare su un progetto di legge che riguardasse la liberazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Si è parlato molto di liberalizzazioni, ma non si parla della liberazione dei cittadini e delle imprese dai vincoli della burocrazia, delle scartoffie, della della presenza del pubblico in attività che dovrebbero essere, invece, lasciate alla libera iniziativa ed al libero esercizio da parte dei privati. Non è un caso che questo disegno di legge abbia una fonte parlamentare non governativa e che - è noto non governativa e che - è noto - sia stato approvato dalla Camera dei deputati non senza parecchi mal di pancia da parte della sinistra radicale e dei

con altrettanti mal di pancia e mugugni da parte della sinistra radicale e dei Verdi, dei quali è noto il carattere statalista e centralista della loro azione politica.

dei cittadini e delle imprese dagli orpelli e dai pesi della pubblica amministrazione? Certamente no. Ricordo che nella passata legislatura sono stati fatti alcuni passi in avanti. avanti. Ad esempio, si è disciplinato diversamente il silenzio-assenso; si è prevista la sostituzione della denuncia di inizio attività ad alcuni tipi di autorizzazione; soprattutto, si è previsto nella legge di semplificazione 2005, della quale sono stato relatore, una norma di delega al Governo delega che è ancora in piedi, perché scadrà alla fine di quest'anno e potrebbe essere eventualmente prorogata - che autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione delle autorizzazioni pubbliche per l'esercizio di attività di impresa. È una delega molto ampia, ma di essa, e riprendo quanto detto all'inizio, non si è mai fatta parola: nessuno ha assunto l'iniziativa; il ministro Bersani, così sensibile ai costi a carico delle imprese, non ha sollecitato i colleghi Ministri competenti ad esercitarla. Si è preferito rincorrere questo mito della liberalizzazione attraverso interventi autorizzativi sul mercato, sulla concorrenza - laddove esistono autorità che avrebbero potuto,

lo approvi in via definitiva. Sarebbe infatti il segnale importante che tutto il Parlamento, nella sua stragrande maggioranza, è sensibile ad un processo di liberazione delle imprese, che in quest'anno e mezzo ha subito un fermo, se non addirittura un arretramento.

anzitutto rassicurare il senatore Pastore che i Verdi non sono assolutamente portatori di un'idea centralista e statalista, anzi, è esattamente il contrario. I Verdi, sono però portatori, questo lo voglio rivendicare anche durante l'esame di questo provvedimento, di norme chiare, precise,

vogliamo che anche l'attività di impresa si possa svolgere secondo regole precise, in particolare, secondo le regole che attengono al governo e alla programmazione del territorio e alla capacità degli enti locali, che poi alla fine sono i soggetti più esposti ai grandi problemi che si verificano nella gestione del territorio e nel rapporto con il mondo delle imprese, i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi diffusi sul territorio. La sfida è sempre questa. La sfida è garantire che queste attività avvengano nel miglior modo possibile, rispettando le regole ed il territorio perché quando si producono danni al territorio e quando si producono danni perché non sono state rispettate le regole non si arreca danno nella situazione specifica, ma in generale, e successivamente è difficile tornare indietro, ripristinare le condizioni

presi dalla fretta e dalla necessità di dimostrare che si sarebbe approvato subito un provvedimento a favore dell'attività d'impresa, non si sia esaminato bene, nel merito e con rigore, il provvedimento. Forse anche sulla spinta dello stesso presentatore originario di questo disegno di legge, l'onorevole Capezzone che, in qualità di Presidente della Commissione

chi sia il presentatore di questo disegno di legge: è un disegno di legge d'iniziativa di un deputato, quindi parlamentare, o anche il Governo ci ha messo del suo, quindi è un provvedimento anche d'iniziativa governativa? Chiaramente, in questa seconda ipotesi, la maggioranza dovrà compiere uno sforzo aggiuntivo per arrivare ad un esame conclusivo e rigoroso

come mai non sono stati presi in seria considerazione le osservazioni, i pareri espressi da alcune Commissioni, in particolare dalle Commissioni 1a e 13a. Dico questo Dico questo perché le Commissioni 1a e 13a a mio parere hanno centrato la questione, hanno fatto in modo che questo ramo del Parlamento

buona che crea lavoro e occupazione, dall'altra garantire regole certe alle quali tutti devono attenersi. Voglio ora ricordare una parte del parere espresso dalla 1a Commissione che ad un certo punto recita: «non è stata accolta la richiesta della 1a Commissione di modifica dell'articolo 9, comma 4, cui era subordinato il parere, peraltro non favorevole bensì semplicemente non ostativo (parere di costituzionalità, ovviamente). La Commissione affari costituzionali ha inoltre osservato che il disegno di legge introduce una rilevante compressione delle autonomie costituzionalmente protette di Regioni e enti locali. Mi sembra questo un tema molto rilevante. Nel parere si legge: «Si segnala pertanto la opportunità di un maggiore coinvolgimento di tali autonomie, in specie per quanto riguarda i profili urbanistici e di gestione del territorio, nonché di tutela ambientale», anche dopo le modifiche apportate in Commissione.

quindi necessario escludere che il semplice rilascio di ricevute possa dare titolo all'avvio delle attività e costituire titolo edilizio». Questo diventa uno stravolgimento delle regole finora vigenti. - «appare non condivisibile il totale esonero da ogni autorizzazione previsto dall'articolo 1, comma 8, in assenza di chiarimenti circa le caratteristiche e l'impatto ambientale delle specifiche attività, cui si applicherebbe l'esonero, svolte nell'area interessata». Inoltre - insiste la Commissione -, «si ritiene necessario prevedere il rigetto delle domande in contrasto con i piani urbanistici, attribuendo in ogni caso ai Comuni, con apposita delibera consiliare, la potestà di individuare e delimitare aree del loro territorio all'interno delle quali, previa approvazione di apposite varianti urbanistiche, possano essere insediate attività conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro, di tutela della pubblica incolumità ». In fondo, questa è la sostanza delle leggi urbanistiche vigenti nel nostro Paese. Il rischio è che con

alla programmazione e alla gestione oculata del territorio, che danno il potere agli enti locali di esercitare quanto previsto dalle norme vigenti. Se passasse un'idea diversa e venisse scardinato questo principio, i Comuni perderebbero perderebbero molta della loro autonomia e della loro forza. I Comuni sono forti quando ci sono regole forti che garantiscono il rispetto di tutte le norme; quando ci sono regole deboli